"Il link apre una nuova finestra"). Comunico che, in data 31 agosto 2013, è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione:* «Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» finestra"). L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione che abbiamo presentato nei mesi scorsi a prima firma del nostro presidente Zanda, e che ci apprestiamo a discutere assieme a quelle di altri Gruppi, riguarda una grande questione nazionale: l'elevato dissesto idrogeologico che vive il nostro Paese. L'Italia, infatti, per le particolari condizioni climatiche e geomorfologiche, è un Paese ad alto rischio geologico ed idraulico, la cui fragilità è sempre più evidente e documentata: i dati forniti sia dal Ministero dell'ambiente che dall'ISPRA ci dicono che nel 2012 sono stati censiti ben 85 eventi di frana principali

A questo preoccupante quadro si aggiunga che nel periodo 2008-2012 abbiamo assistito ad un aumento delle vittime degli eventi alluvionali, con un'interruzione del precedente *trend* in diminuzione, negli anni 2001-2007, dovuta anche a mutate condizioni climatiche a cui il continente europeo è sottoposto. Si stima che la popolazione esposta ad alluvioni ed altri eventi del genere ammonti attualmente a oltre 6.100.000 abitanti. Che il dissesto idrogeologico sia ormai una vera e propria priorità nazionale è dimostrato anche dal fatto che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presentato già nei primi cento giorni di Governo ben due disegni di legge in materia, certamente apprezzabili, il primo per il contenimento del consumo e per il riuso del suolo, il secondo sulle demolizioni nelle aree a dissesto idrogeologico: questo - ne siamo convinti - di una rinnovata e decisiva attenzione verso le tematiche ambientali e ad un fenomeno specifico che è cresciuto a ritmi impressionanti. Sempre secondo i dati dell'ISPRA, in Italia sono stati consumati, in media, 7 metri quadri al secondo di suolo per oltre 50 anni, con un picco di 10 metri quadri negli anni Novanta e un valore odierno di 8 metri quadri. In termini assoluti sono stati persi in modo irreversibile ben 20.500 chilometri quadrati. Si è assistito cioè, negli ultimi decenni, ad una crescita continua dell'urbanizzazione, a volte incontrollata, al proliferare di interventi artificiali su corsi d'acqua, fiumare e canali, e alla sottrazione di aree allagabili e di aree libere, agricole e boschive: si tratta di aree che rappresentano presidi essenziali per la tenuta del territorio italiano, di cui si paga un prezzo altissimo ogni qualvolta, sul Paese, si abbattono eventi atmosferici particolarmente intensi. Gli eventi alluvionali che hanno colpito anche nell'ultimo anno i territori dell'Emilia-Romagna e della Liguria (segnalati fra l'altro dall'apposita mozione n. 21) i dissesti dei territori appenninici che ne sono seguiti, nonché quelli che hanno colpito ripetutamente altre Regioni, dimostrano quanto il problema del dissesto idrogeologico non sia più catalogabile nella logica dell'emergenza, sia a causa della frequenza degli eventi sia per la gravità delle conseguenze sui territori coinvolti. in esame, onorevoli colleghi, intendiamo in primo luogo mettere in luce come occorra passare dalla logica dell'emergenza a quella della prevenzione nella gestione del territorio.

di non occupazione o ripristino delle aree destinate all'espansione naturale dei corsi d'acqua, di minimizzazione del rischio e di misure di adattamento al rischio residuo. È innegabile che nella gestione delle risorse pubbliche per la tutela dell'ambiente si evidenzia un *deficit* di pianificazione e programmazione con una spesa improduttiva e e molte volte dirottata su altre finalità: uno studio della CGIA di Mestre ha indicato che solo l'l,l per cento delle imposte «ecologiche» sull'energia, sui trasporti e sulle attività inquinanti, pagate dai cittadini allo Stato e agli enti locali, è destinato alla protezione dell'ambiente. Più in generale, occorre sottolineare come le politiche di gestione del territorio continuano a destinare la gran parte delle risorse disponibili all'emergenza, anziché a un'effettiva opera di prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Questo rapporto va cambiato e, analogamente al principio che sovrintende al pagamento di alcuni tributi o tasse come quella sui rifiuti (cioè chi inquina paga), dobbiamo lavorare per una fiscalità ambientale che premi i cittadini e le imprese virtuose e penalizzi chi non lo è per investire sul territorio, che rappresenta il valore aggiunto più importante di qualsiasi sistema economico e sociale. Tra il 1999 e il 2008 sono stati impiegati 58 miliardi di euro per la difesa del suolo, la riduzione dell'inquinamento e l'assetto idrogeologico, ma di questi oltre il 50 è stato assorbito dalle spese di parte corrente e solo 26 miliardi di euro sono stati destinati a investimenti per la prevenzione dei rischi. Gli stanziamenti ordinari riguardanti la difesa del suolo e il rischio idrogeologico degli ultimi pesanti riduzioni di risorse, facendo venir meno la certezza di poter disporre degli stanziamenti necessari a politiche di prevenzione, che hanno bisogno di continuità per poter essere efficaci e registrano, nei nei fatti, uno spostamento delle modalità di finanziamento verso la gestione straordinaria. Oltre al tema delle risorse, è necessario mettere mano con decisione all'infrastrutturazione istituzionale nel campo delle politiche per la difesa del suolo. La maggiore criticità oggi riscontrabile è, infatti, dovuta al mancato completamento del riassetto del sistema di *governance* e a una frammentazione e sovrapposizione di competenze tra diversi soggetti e strumenti A livello nazionale si sconta, necessariamente, la mancanza di una regia unitaria che coordini le diverse azioni sulla difesa del suolo e la gestione della risorsa idrica. Nella mozione indichiamo come il sistema di gestione proposto per la difesa del suolo, la tutela delle acque e i servizi idrici vada profondamente cambiato, essendo incapace di coordinare sinergicamente competenze, ruoli, responsabilità e poteri che già ci sono. Chiediamo perciò al Governo un cambio di passo sul tema della *governance* e di aderire alla strategia europea in materia di difesa del suolo, che si fonda sul cambiamento del modello di sviluppo: scelte di destinazione d'uso del territorio, ricostruzione ecologica dei corsi d'acqua, agricoltura come cura e presidio del territorio, analisi economica nei processi decisionali, politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, partecipazione dei cittadini nella ricerca di scelte condivise. Oggi la maggior parte degli interventi finalizzati alla difesa del suolo è costituita da interventi strutturali di difesa passiva, che in termini di costo ed efficacia si sono rivelati non pienamente soddisfacenti. Al contrario, occorre puntare sulle attività di carattere preventivo, che pongano l'enfasi sul valore delle regole di uso del suolo, sul monitoraggio delle situazioni di rischio e sul grado di conoscenza e consapevolezza delle popolazioni di esposizione al rischio di un territorio. Presupposto essenziale per il passaggio da una logica emergenziale a una basata sulla prevenzione è pertanto la predisposizione di un sistema di finanziamento adeguato, oculato e certo. Da questo punto di vista è apprezzabile la volontà da parte del Ministero dell'ambiente di istituire, di concerto con gli enti territoriali, un fondo nazionale per la difesa del suolo e la riduzione del rischio del rischio idrogeologico. Occorre individuare un meccanismo finanziario in grado di generare risorse certe ogni anno, per finanziare gli interventi di riqualificazione, garantendo una disponibilità finanziaria sicura, che permetta di programmare la spesa e avviare il lungo percorso di adattamento del territorio italiano verso condizioni di maggiore naturalità e maggiore sicurezza. È necessario, infine, togliere dalle maglie strette e vincolanti del Patto di stabilità interno le spese e gli interventi attuabili dagli enti pubblici in questo settore, attraverso un piano straordinario di manutenzione diffusa del territorio e dei corsi d'acqua, fatto di mille piccole opere, e anche della sperimentazione di progetti che coinvolgano, nella manutenzione ordinaria di aree verdi, boschive e fluviali, i lavoratori temporaneamente beneficiari di ammortizzatori sociali o i detenuti. Un piano che peraltro coinvolga il sistema delle autonomie locali e che rechi forme di incentivazione della partecipazione attiva della popolazione singola o associata, come ad esempio i contratti di fiume. Con questa mozione intendiamo perciò richiamare ad un nuovo e più incisivo impegno il Parlamento e il Governo, anche alla luce dei deludenti risultati registrati negli ultimi anni individuare soluzioni tempestive e avanzate per fronteggiare il ripetersi di episodi calamitosi ed emergenziali. Abbiamo la necessita impellente di un cambio di passo istituzionale e culturale e l'impostazione avviata dal nuovo Ministero ci fa ben sperare. La nuova legge di stabilità per il 2014 deve essere il banco di prova per misurare la coerenza tra il dire e il fare nell'interesse del Paese e del territorio, spostando certo nuove risorse su questa priorità nazionale, ma soprattutto indicando l'avvio di una nuova stagione di politiche pubbliche. Il Partito Democratico è pronto a sostenere e a vincere questa sfida, assieme a tutte le forze politiche che in quest'Aula hanno a cuore come noi lo sviluppo sostenibile e inclusivo del nostro Paese e delle sue risorse naturali

la mozione che abbiamo presentato come Gruppo Misto, componente SEL, sul dissesto idrogeologico è stata uno dei primi atti che abbiamo voluto compiere, perché riteniamo che non sia più rinviabile un'assunzione di responsabilità e un cambio deciso delle strategie del nostro Paese in questo campo. I dati degli ultimi anni ci dicono che la fragilità strutturale del nostro Paese si è ulteriormente aggravata. I sempre più frequenti fenomeni alluvionali e calamitosi che colpiscono l'Italia non solo mettono in luce con drammaticità l'estrema fragilità del nostro territorio, ma ci dicono ormai con chiarezza che non sono più procrastinabili un progetto e una strategia complessiva di messa in sicurezza. Tutto ciò accompagnato ad una politica innovativa e di svolta sulla pianificazione urbanistica del nostro territorio. A questi dati sui sempre più frequenti fenomeni alluvionali si deve aggiungere, colleghi, il crescente grado di erosione costiera, che ormai interessa oltre 540 chilometri lineari lineari dei litorali italiani, in cui sono direttamente coinvolti i beni più preziosi del nostro sistema Italia: i sistemi paesaggistici e il territorio. I dati sulle

dati ci dicono, appunto, che stiamo parlando di una cementificazione assolutamente legale e questo non può che essere imputato a delle politiche di pianificazione urbanistica - qualora ci siano pianificazione o scelte edilizie nei nostri territori - che stanno mettendo sempre più a rischio il bene Paese e quello che noi riteniamo un bene comune, ossia il suolo. Questi dati ci dicono anche che, gli effetti dei cambiamenti climatici in atto sono tali per cui gli eventi estremi in Italia hanno subito un aumento esponenziale, passando da uno circa ogni 15 anni (prima degli anni Novanta) a 4‑5 all'anno. La questione dei cambiamenti climatici (che, ahimè, purtroppo, continua ad essere ampiamente sottovalutata) non può rimanere estranea alla discussione che facciamo oggi sul dissesto idrogeologico. Vorrei qui richiamare gli ultimi dati che sono stati pubblicati su autorevoli

da questo punto di vista, dobbiamo aspettarci che questi eventi estremi possano aumentare sempre di più. A fronte di questa situazione così pesante, sappiamo anche che nel nostro Paese sono mancati una politica nazionale seria, un coordinamento delle azioni e una strategia che ponessero in modo strutturale la priorità della messa in sicurezza del nostro territorio. D'altronde, basta vedere i dati economici per capire come sono state spese le risorse Vorrei qui ricordare che il rapporto tra risorse per la prevenzione e risorse per l'emergenza è di 1 a 100: a fronte di 2 miliardi di euro spesi in prevenzione, per la messa in sicurezza e per gli interventi per la salvaguardia del territorio, abbiamo una spesa per l'emergenza che è

il 10 per cento della superficie nazionale del Paese è ad alta criticità idrogeologica e sono oltre 6.600 i Comuni interessati: quindi, stiamo parlando davvero di una situazione molto seria e grave. A questo dobbiamo aggiungere altri dati che sono strettamente connessi. Non possiamo oggi fare l'errore di affrontare la questione del dissesto idrogeologico senza affrontare parimenti, con la stessa fermezza, la questione del consumo del suolo nel nostro Paese: le due questioni, infatti, come molti di voi sanno perfettamente, sono strettamente connesse. I dati del consumo del suolo nel nostro Paese sono sono assolutamente spaventosi e allarmanti. Una ricerca eseguita qualche tempo fa dal WWF Italia con l'Università dell'Aquila ha fatto emergere dati che devono far riflettere tutti. Dal 1956 al 2001 la superficie urbanizzata del nostro Paese è aumentata del 500 per cento; tra il 1990 e il 2005 si è stati capaci di trasformare oltre 3 milioni e mezzo di ettari, cioè una superficie grande quasi quanto il Lazio e l'Abruzzo messi insieme.

non ci danno segnali in controtendenza, ma di ulteriore incremento. Noi non possiamo più permetterci per la sicurezza del Paese e per la tutela del del territorio - che, torno a ripetere, è un bene comune - di continuare a consumare il suolo con questi ritmi. Bisognerà arrivare ad una moratoria; il Governo ha approvato un disegno di legge ed altri disegni di legge sono stati presentati per lo *stop* al consumo del suolo. Bisogna assolutamente invertire la tendenza. Oltre a ciò, in questi anni, proprio perché è mancata, a nostro avviso, la consapevolezza della priorità dell'intervento sul dissesto idrogeologico e della messa in sicurezza, sono state fatte politiche di *governance* molto disordinate, in contrasto le une con le altre. Non vi è stata un'omogeneità di interventi.

ormai quasi da tutti completamente sbagliati. Anche su questo bisognerà cambiare completamente la strategia. La nostra mozione in breve chiede - il Ministro dell'ambiente ha annunciato questo fondo - in raccordo con le Regioni un vero e proprio piano pluriennale per la difesa del suolo

perché, tra l'altro, intervenire e considerare la prima opera prioritaria per il Paese la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico e la difesa del suolo significa anche creare economia

l'altra proposta che facciamo è quella di un piano giovani, per far sì che si intervenga con una serie di opere di manutenzione nella difesa del suolo. *(Applausi della

fa il punto sulla gravità della problematica. Il nostro Paese è caratterizzato da una ricchezza di corsi d'acqua per la presenza massiccia di aree montuose, ove il dissesto idrogeologico è un fenomeno ricorrente e fortemente legato anche alla giovane età geologica del nostro territorio. Fenomeni naturali quali i processi erosivi delle coste, le esondazioni, le frane e le alluvioni, insieme ai terremoti e agli incendi, concorrono a determinare ingenti danni umani, materiali e ambientali. L'intervento antropico sul territorio ha, in diversi casi, aumentato notevolmente l'impatto di tali eventi, accelerando fenomeni distruttivi e rendendo il territorio ancor più vulnerabile. La corsa alla cementificazione, il consumo non regolato del territorio, i disboscamenti, l'abusivismo edilizio, la dissipazione dissennata delle risorse, associati ai tagli dei fondi destinati alla sicurezza ambientale, sono tutti fattori che messi insieme accrescono strutturalmente la gravità della situazione. Dal 1960 al 2012 si sono verificati sul territorio nazionale 1.453 eventi tra frane e inondazioni, con 2.836 feriti e 4.132 morti. Sembra un bollettino di guerra e dà il senso della gravità della situazione.

il Paese si è dotato di un sistema di allerta per il rischio idrogeologico, la cui gestione è assicurata dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e da una rete che coinvolge gli enti locali. In realtà, la spesa annua - calcolata in oltre 300 milioni di euro - per attuare strategie di intervento straordinario volte a ripristinare lo *status quo ante* dei luoghi e delle cose, pesa in maniera inesorabile sui bilanci pubblici e consente di ripianare solo un terzo dei danni registrati. Nel 2009 il CIPE assegnò un miliardo di euro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, che avrebbe dovuto innestarsi in un piano straordinario di 2,5 miliardi di euro per gli investimenti più urgenti per le piccole e medie opere dirette a rimuovere le situazioni di alto rischio idrogeologico, messo a punto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; dopo anni di incertezze, lentezze, inerzie finanziarie, tale finanziamento è stato tagliato dalla legge di stabilità per il 2011 e quindi non è utilizzabile. Pertanto, noi con questa mozione vorremmo in primo luogo impegnare il Governo a dare esecuzione immediata al Piano straordinario per la difesa del suolo avendo messo in campo 2,5 miliardi di euro fra fondi statali e cofinanziamenti regionali potrebbe anche adire a risorse europee; ad assumere iniziative di competenza affinché sia previsto nel bilancio dello Stato uno stanziamento annuale aggiuntivo destinato alla manutenzione ordinaria del territorio e da destinare sulla base delle decisioni della Conferenza Stato-Regioni-autonomie locali; prevedere specifiche norme per l'applicazione, laddove possibile, dei criteri di ingegneria naturalistica agli interventi di prevenzione del sistema idrogeologico; attuare decise politiche di riassetto dei suoli, nel rispetto dei limiti delle competenze *ex* articolo 117 della Costituzione in materia di tutela ambientale e dell'ecosistema, attraverso iniziative e provvedimenti indirizzati alla promozione di strategie per la messa in sicurezza dei territori

supportando i sindaci in una capillare e semplificata campagna di informazione ai cittadini relativamente ai comportamenti di autoprotezione, nonché in termini di conoscenza dell'esposizione al rischio delle infrastrutture pubbliche e private, secondo quanto previsto dai piani comunali di protezione civile, evitare la sovrapposizione di competenze tra i soggetti coinvolti negli interventi, sostenendo l'identificazione nel Dipartimento della protezione civile dell'organismo di coordinamento, che svolge imprescindibili funzioni di raccordo tra i vari soggetti interessati ai diversi livelli di competenza nell'ambito delle attività di previsione, prevenzione e gestione dell'emergenza, nel rispetto di quanto disposto disposto dalla normativa vigente in materia di Protezione civile e dalle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri. Per quanto riguarda invece l'ordinarietà, della quale dovremmo interessarci, si potrebbero valorizzare, per esempio, le competenze dei consorzi di bonifica, che sono distribuiti su tutto il territorio nazionale e che hanno, appunto, competenze acquisite negli anni sulla prevenzione del dissesto idrogeologico. contrastare iniziative legislative volte ad introdurre forme di condono edilizio, ovvero la proroga di termini per condoni già concessi negli anni passati, ove possano aumentare il rischio idrogeologico; definire parametri coerenti per consentire alle imprese alluvionate di accedere ad una disciplina fiscale di favore o a forme di finanziamenti agevolati, con l'esenzione dal pagamento di quote capitali e interessi e/o attraverso iniziative di rinuncia alla riscossione dei tributi locali o della sospensione, a livello nazionale, del pagamento dell'Irpef.

Signor Presidente, onorevoli senatori, l'argomento che il Senato sta trattando riguarda una problematica complessa e multidisciplinare rispetto alla quale è necessario assumere misure in grado di dare risposte alle esigenze di prevenzione, alle necessità di manutenzione ordinaria ed alle richieste di intervento urgente. Data la vastità del tema è possibile, ovviamente, fornire solo qualche spunto. Fenomeni di natura alluvionale e calamitosa interessano da decenni gran parte del nostro territorio nazionale. Sulla base delle classificazioni elaborate dal Ministero dell'ambiente è noto che più del 10 per cento della superficie dell'intero Paese è inquadrato come area ad alta criticità idrogeologica. Ma il dato che meglio evidenzia la problematica di cui si tratta è che oltre l'80 per cento delle comunità locali è potenzialmente interessato da fenomeni di rischio idrogeologico. La fragilità del territorio italiano ha comportato pesanti conseguenze anche sotto il profilo della perdita di vite umane. Si pensi infatti che oltre 150 sono state le vittime causate dai soli eventi alluvionali dall'inizio del nuovo secolo e quasi 800 le vite stroncate da analoghi fenomeni accaduti subito dopo i già tragici fatti del 1966 e sino all'anno 2000. Il numero dei morti sale vertiginosamente se si riporta alla memoria l'immane tragedia del Vajont (di cui quest'anno ricorre il 50° anniversario), la tragedia di Stava ed altre ancora connesse con una scarsa conoscenza del territorio e con un atteggiamento tracotante dell'ingegneria e della geotecnica. I fenomeni legati all'instabilità idrogeologica hanno altresì causato negli anni enormi danni alle attività socio-economiche e produttive, interessando molte aree del nostro Paese. A fronte di questi drammatici elementi è necessario richiamare recenti studi che hanno illustrato come la pericolosità idraulica e geologica del territorio italiano sia sensibilmente aumentata negli ultimi anni e con essa la vulnerabilità del territorio stesso, ciò anche a causa di discutibili scelte di pianificazione nell'uso del suolo; basti citare il caso della formazione di insediamenti, abitativi e produttivi, realizzati in assenza di qualunque pianificazione per il riassetto idraulico del territorio. L'esposizione di molte aree al pericolo di inondazione altro non è che il frutto di una cattiva gestione della gerarchia degli strumenti di programmazione e pianificazione dell'uso del territorio e, nello specifico, un'anteposizione dell'urbanizzazione alle esigenze idrauliche. Per tale ragione è bene comprendere che la problematica in esame si caratterizza per essere attraversata da profili di multidisciplinarità assai marcati, come evidenziano le più recenti leggi urbanistiche regionali in termini positivi e virtuosi. Ciò significa che la predisposizione di interventi finalizzati alla mitigazione dei fenomeni calamitosi di origine idrogeologica richiede innanzitutto un'attenzione competente verso tutti gli ambiti coinvolti, che si possono sinteticamente riassumere nella formula della necessaria convivenza tra l'obiettivo della tutela delle attività antropiche con la conoscenza e la valorizzazione dell'ambiente nel quale esse si inseriscono. In secondo luogo, è richiesto un convinto passaggio ad un approccio di sistema che abbia il fine di consentire una costante e diretta conoscenza dei dati e il loro utilizzo finalizzato sia alla prevenzione sia alla risposta alle esigenze del presente. I punti fondamentali della mozione riguardano: un'azione di coordinamento attraverso la quale superare l'attuale frammentazione e sovrapposizione delle competenze; la promozione di interventi di semplificazione nell'ambito delle procedure amministrative e autorizzative; il rilancio di un vero e proprio sistema della conoscenza che miri all'acquisizione e allo scambio su scala nazionale delle informazioni e dei dati inerenti i fenomeni da monitorare e mitigare la promozione di una necessaria complementarietà tra le attività di prevenzione, gli interventi di gestione ordinaria e la manutenzione straordinaria ed urgente, elementi essenziali per la gestione del territorio. La mozione, dunque, intende impegnare il Governo essenzialmente sulle seguenti attività. Innanzi tutto, si chiede un forte intervento di semplificazione dell'attuale sistema di *governance*, un sistema che è stato progressivamente costruito con provvedimenti *ad hoc* e che tuttavia ha mostrato numerosi limiti operativi a causa della presenza di un eccessivo numero di attori; se, infatti, sotto il profilo teorico il ricorso alla logica delle deleghe può rispondere all'obiettivo di avvicinare al territorio la gestione delle problematiche in materia ambientale, da un punto di vista pratico tale sistema è invece esposto al depotenziamento della filiera delle responsabilità. Si chiede, perciò, al Governo di intervenire per confermare la strutturazione su base regionale o subregionale, formulando l'indirizzo di una chiara semplificazione, naturalmente salvaguardando e valorizzando le realtà amministrative e gestionali che hanno dimostrato nel tempo la propria insopprimibile efficacia. Una tale impostazione richiede evidentemente la necessità di ottimizzare tali soggetti in termini di strumenti, risorse umane ed attribuzione delle competenze, di modo che essi possano agire con efficacia e prontezza tanto - come già evidenziato - nella pianificazione quanto nella gestione delle urgenze. la mozione si chiede altresì che si intervenga - sempre in una logica di sistema - al fine di ridurre il distacco tra la conoscenza prodotta dalla ricerca e le applicazioni utili per la società civile. La gravità delle statistiche richiamate in premessa richiede, infatti, che si usi largamente delle attuali disponibilità legate al sapere e all'informare, al prevedere e al gestire, in modo che nella difesa idrogeologica e nella gestione dei rischi siano assorbite le opportunità operative connesse con l'applicazione delle delle nuove tecnologie. Si chiede perciò al Governo un impegno fattivo al fine di supportare le attività di ricerca e, ancor più, di scambio delle informazioni raccolte sul territorio nazionale, nella logica già molto diffusa nell'ambito informatico del riuso di pratiche di buona tecnica, di pratiche di monitoraggio e di pratiche di allerta e pronto intervento. È infatti vero che per lo studio, la prevenzione e la protezione civile, connessi con i problemi del rischio idrogeologico, sono disponibili oggi strumenti di previsione formidabili, che è indispensabile far entrare nell'utilizzo quotidiano degli enti; mi riferisco ai modelli matematici idrologico-idraulici, alla modellazione numerica, alla raccolta sistematica di dati e al monitoraggio di parametri ambientali e climatici da attuarsi anche attraverso il consolidamento delle attività delle ARPA, insieme ad una sistematica diffusione e condivisione nazionale è vero che ogni singolo bacino idrografico richiede di essere studiato attraverso specifiche attività di raccolta dati, è altrettanto vero che l'inserimento nella rete dei sistemi informativi territoriali delle singole esperienze locali può consentire un più rapido e corretto scambio utile alla pianificazione anche in sede nazionale, nella logica dell'estensione degli obiettivi dell'Agenda digitale anche ai temi della gestione dei rischi idrogeologici. Quanto evidenziato richiede una conseguente attività di semplificazione degli *iter* amministrativi e autorizzativi, con l'obiettivo primario di garantire costi e tempi certi connessi con le attività richieste. Si è sin qui formulato l'indirizzo che gran parte degli sforzi debba essere orientata alla prevenzione dei fenomeni connessi con il rischio idrogeologico, tuttavia non è bene che tale impostazione induca alle logiche dell'immobilismo di fronte agli interventi che già oggi assumono caratteri della massima urgenza. La prevenzione è necessaria affinché si superino e non si ripetano quegli errori che hanno condotto alla situazione attuale, ma la prevenzione nulla può di fronte alle problematiche in essere che chiedono risposte immediate. Peraltro, il territorio evolve non solo in ragione degli interventi antropici, ma anche per fattori naturali, ed è quindi necessario guardare all'equilibrio uomo-ambiente come a un obiettivo flessibile, dinamico e non ideologico. Infine, si riporta l'attenzione su tre tipologie di intervento per la cui attuazione si formula un preciso indirizzo. In primo luogo, si chiede di poter pervenire, d'intesa con i proprietari e gestori degli invasi, ad un migliore monitoraggio dello stato delle grandi dighe presenti sul territorio nazionale, veri e propri volumi utili al contenimento delle piene nei tratti di valle, attraverso un'attività di mantenimento della capacità di invaso dei serbatoi, da attuarsi sia con una programmazione delle attività di sghiaiamento, sia con una revisione dei disciplinari di esercizio. In secondo luogo, si chiede al Governo di dare supporto in termini di semplificazione alla realizzazione delle casse di espansione, che rappresentano una risposta di relativamente semplice attuazione alle gravi crisi idrogeologiche

formazione delle maestranze, che siano in grado di gestire un sistema adeguato e costante degli alvei. In definitiva, si tratta di un insieme di azioni che permettano di cogliere appieno connesse all'uso delle moderne tecnologie e metodologie, di adeguare la legislazione al fare concreto e di favorire, perciò, l'incremento della sicurezza delle famiglie, delle imprese e delle infrastrutture, nella logica del miglioramento della qualità della vita della società italiana, alla luce di un equilibrato rapporto con l'ambiente e il territorio. Ha facoltà di parlare il senatore Arrigoni per illustrare la mozione n. 137. in via preventiva con mezzi concreti e con risorse finanziarie stabili, che regolarmente devono essere stanziate dal bilancio dello Stato, sono palesi e noti sia alle istituzione sia ai cittadini, che attendono interventi veri, che vadano oltre le discussioni nelle Aule parlamentari.

Purtroppo le avversità atmosferiche non accadono con frequenza costante nel tempo o con fattori di incidenza che possano preannunciarle. L'unica sicurezza che abbiamo è che i disastri che si manifestano oggi a seguito di fenomeni meteorologici eccezionali sono inscindibilmente collegati alla vulnerabilità e alla fragilità del territorio e alla struttura idraulica e geologica del terreno. Perché ultimamente i disastri da alluvioni e frane sono sempre più frequenti, sempre più intensi e sempre più catastrofici? Da una parte attraversiamo un periodo di cambiamenti climatici, che non sono necessariamente collegati al riscaldamento del globo si tratta comunque di cambiamenti climatici del nostro periodo storico, che in ogni caso sono collegati anche alla deforestazione o alle trasformazioni territoriali a livello globale. D'altra parte, l'aumento dei disastri è senz'altro dovuto al non corretto uso del suolo, sia per la cattiva amministrazione del territorio sia per il suo abbandono, lo spopolamento della montagna e dei piccoli centri e l'incuria del territorio, legata alla perdita del contatto con lo stesso. I casi di abusivismo edilizio sono i primi della lista nel provocare i disastri annunciati. La costruzione abusiva di edifici ai margini, se non persino nell'alveo dei torrenti e dei fiumi o su un terreno franoso,

Spesso sono gli stessi piani regolatori ad essere stravolti da mille compromessi, che perseguono interessi di parte e non la compatibilità con le caratteristiche ambientali del territorio. Il disastro avvenuto a Messina è l'esempio lampante della cattiva amministrazione del territorio: il rilascio di autorizzazioni edilizie nel letto di un torrente si pone al di fuori di ogni logica di buon governo. Cosa fare dunque per il futuro? In Europa, come è già avvenuto in America, si parla ormai di strategia di adattamento, intesa non come adattarsi agli eventi, ma come prevenzione dei danni futuri. La strategia di adattamento è una strategia di mitigazione del rischio che agisce sulla prevenzione degli effetti negativi e dei danni provocati dai cambiamenti climatici, indipendentemente dalle misure di contenimento delle emissioni stabilite a livello mondiale dai vari protocolli e normative (protocollo di Kyoto, direttive sulle emissioni, il contenimento energetico ed altre ancora). La strategia di adattamento ai rischi compete al singolo Paese, che l'attua con strumenti e programmi propri; si tratta di una cornice di riferimento alle scelte e agli interventi di gestione del rischio di competenza delle autonomie locali e regionali. Gli altri Paesi europei, sollecitati da iniziative della Commissione europea, stanno avviando proprie strategie nazionali di adattamento; sarebbe ora che anche il nostro Paese seguisse tali strategie.

stamani, come quelle presentate ed approvate lo scorso 26 giugno alla Camera dei deputati, rappresentano un primo passo, ovviamente con diverse sensibilità, verso un cambiamento della strategia sin qui adottata per affrontare il tema della difesa del suolo e del rischio idrogeologico. La mozione presentata dal Gruppo Lega Nord impegna in particolare il Governo affinché si privilegi

per facilitare procedure meno farraginose, come invece quelle attuali e vigenti, in ordine all'efficacia degli interventi; di predisporre e attivare un programma organico di interventi e di prevedere nel bilancio dello Stato uno stanziamento annuale stabile destinato alla manutenzione del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico; di coinvolgere maggiormente gli enti locali e le Regioni per l'individuazione, la programmazione e l'attuazione degli interventi. Voglio sottolineare, come sia importante e fondamentale il ruolo dei sindaci ed anche dei semplici consiglieri comunali, che non percepiscono forse nulla o un semplice gettone di presenza di circa 10 o 20 euro al mese, che magari devolvono alla loro comunità, e che quotidianamente percorrono in lungo e in largo il loro territorio, gli alvei dei fiumi, i monti e le colline, segnalando i pericoli e mettendo a disposizione il proprio tempo, insieme ai volontari del territorio, per fare opere di prevenzione e sistemazione dei danni;

Presidente, oggi parliamo di dissesto idrogeologico e spesso abbiamo sentito dire che l'Italia è un Paese ad alto rischio;

l'errore che commettiamo è quello di confondere le aree a criticità con le aree a rischio. Le aree a criticità sono sostanzialmente la somma delle aree pericolose e delle aree a rischio. L'area pericolosa è un'area dove può avvenire una frana, ma non c'è un elemento vulnerabile che viene colpito dalla frana. Quindi facciamo un errore ed una sovrapposizione erronea,

aree a rischio a questo punto si tratta di un rischio importante, perché il rischio è una moltiplicazione: è il prodotto della pericolosità per il valore esposto (cioè quanto vale il bene esposto a rischio moltiplicato la vulnerabilità, cioè il grado di quanto si danneggia il bene).

Quindi, quando parliamo di rischio dobbiamo stare attenti. Ovviamente, il problema è molto grave: è un problema molto sentito, e noi siamo molto sensibili a tale

siamo ancora con le autorità di bacino. Questi sono i controsensi che viviamo noi operatori dell'ingegneria e, in questa fase, noi operatori della legge. Il Piano per l'assetto idrogeologico, che è lo stralcio del Piano di bacino, rappresenta tutte le situazioni e individua tutte le zone dove c'è pericolosità. Questa pianificazione si sovrappone ai vari PTCP (piani territoriali di coordinamento provinciale) e ai piani regolatori. Noi sappiamo dunque in maniera specifica e precisa dove sussiste il rischio, quali sono le zone, le aree, le case, gli insediamenti.

si potrà costruire. Bisogna però essere molto chiari: è impossibile costruire qualcosa in un'area dove sussiste una pericolosità. Quindi, dobbiamo dare valore di nullità a qualsiasi atto che viene rilasciato. Tutto ciò nasce dalla mitica legge n.183

Ma come si fa a gestire una cosa del genere? Che sia un unico distretto il bacino del Po mi pare logico, ma nell'Italia meridionale ci sono tanti piccoli bacini. Un signore che deve fare un intervento a Reggio Calabria deve andare a Caserta per farsi rilasciare un'autorizzazione: ma vi pare una cosa logica? Che efficacia c'è in tutto questo?

Signora Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, considero la discussione sul tema del dissesto un appello al Governo e insieme a tutte le istituzioni che hanno, a varo titolo, competenze sulla tenuta e sulla sicurezza del territorio. È adesso il momento di una forte discontinuità; adesso, nel mezzo di una recessione senza precedenti per il nostro Paese, occorre avere il coraggio di un'inversione di rotta, di una nuova cultura - com'è stato detto bene dal collega Vaccari - e di un cambio di passo, un approccio completamente ribaltato: manutenzione del territorio come pratica ordinaria e non continua rincorsa all'ultima emergenza; tramutare la straordinarietà e la logica delle grandi opere in migliaia di piccole intelligenti manutenzioni, questa è la rivoluzione culturale che è poi anche rivoluzione economico-finanziaria: piccoli e diffusi interventi di qualità, che sostengono, prevedono o rafforzano preventivamente, rendono consapevoli e responsabili le persone che fanno vivere, lì sul loro territorio, le piccole e medie imprese. Quindi, Quindi, manutenzione come attività continuativa e diffusa per ripristinare, migliorare e garantire la piena funzionalità del territorio. ribaltare l'approccio: riuso e rigenerazione di terreni e di immobili; riqualificazioni, più che continue e nuove costruzioni, che consumano suolo pur non avendo una domanda abitativa corrispondente, o chilometri di capannoni, ormai inutilizzati, che sono rimasti scheletri di cemento senza imprese dentro. Questo è di una miopia di programmazione che ha continuato a coltivare l'idea di uno sviluppo basato sui metri cubi e non sulle competitività delle conoscenze e delle tecnologie e le infrastrutture immateriali. È così: si è costruito troppo e ovunque, si è andati a quantità e non a qualità. In quarant' anni ci siamo consumati un'estensione di terreno pari a due grandi Regioni; in poco più di cinquant'anni si è quasi triplicato il consumo di suolo. È urgente invertire la rotta e il Governo deve guidare questo nuovo corso, sapendo che non solo di cambiamento del pubblico si tratta, non solo di leggi e di decreti si tratta, ma di diversi soggetti coinvolti in questo processo e quindi di un mutamento culturale ben più ampio. esempio, nel settore delle costruzioni siamo ancora dentro alla logica dell'azione ad effetto e guadagno immediato, in una catena delle convenienze. Il valore generato dalla rendita immobiliare, infatti, ha premiato e prodotto una serie di convenienze per più soggetti: per la proprietà del terreno, per posizionamento territoriale o contesto urbano; per l'operatore immobiliare, con mutamento facile di destinazione d'uso; per l'investitore, cittadino o società, con il moltiplicarsi del valore dell'immobile nel tempo (non dimentichiamo che per anni la proprietà immobiliare ha rappresentato praticamente l'unico strumento di garanzia per l'accesso al credito e l'indicatore fondamentale di misurazione per l'ente pubblico, fruitore degli oneri di urbanizzazione, una delle entrate determinanti per i Comuni; per la finanza e il sistema bancario, per i consistenti rendimenti provenienti dall'intero ciclo finanziato a debito, e per parti importanti del mondo delle professioni. Questo modello di programmazione negoziata non può essere perpetuato oltre. È cambiato radicalmente, in pochi anni, il contesto: finita la disponibilità di terreno*,* finito il continuo aumento di rendita di rivalutazione, ridotta la fiscalità agevolata, ridotte drasticamente le fonti finanziarie a debito. In compenso, si è reso evidente il costo ambientale prodotto in questi anni, in termini di crescita di vulnerabilità del nostro territorio, grazie ad un'impermeabilizzazione progressiva del terreno, che ha ampliato fortemente gli impatti delle emergenze e degli eventi climatici. Occorre allora avere il coraggio di passare da questa catena delle convenienze ad a una nuova catena di valori a beneficio multiplo, che guardi non solo all'immediato, ma a qualche generazione in avanti;

che riesca a intravedere una vera e propria economia basata sulla cura del territorio e non sulla «rapina e fuga»; una visione che consideri le aree rurali non territori di risulta dell'urbano, ma luoghi di elaborazione di una nuova qualità dello sviluppo che possa rispondere alle criticità contemporanee, come l'inquinamento, il dissesto, l'omologazione, l'anonimato e la generalizzazione. Entrare in una visione diversa significa vedere nell'agricoltura e nei suoi operatori una grande opportunità: riconoscere un nuovo ruolo agli agricoltori, trattenere in montagna i giovani che possono fare impresa agricola, vuol dire modificare l'approccio tra pubblico e settore agricolo. Nonostante le normative comunitarie da tempo abbiano sancito con la multifunzionalità questo ruolo, le risorse pubbliche trasferite agli operatori privati, in particolare alle aziende agricole, assumono ancora oggi la forma del contributo: vengono cioè trasferite a titolo di aiuti al reddito in base ai principi di disaccoppiamento ed ecocondizionalità introdotti dalle normative europee. Credo sia invece decisivo riportare questo scambio di utilità nella veste del contratto con cui la collettività acquista servizi ambientali da agricoltori pienamente investiti da questo ruolo. La ridotta disponibilità di risorse economiche attivabili e la necessità di migliorare l'efficacia della spesa deve essere accompagnata da un riordino complessivo delle logiche che governano l'erogazione di fondi pubblici programmazioni dedicate, specifiche per i territori. Occorrono una programmazione convincente e risorse certe, soprattutto certe: mi azzardo a dire anche poche risorse ma certe, costanti e programmabili. Questo ci può far voltar pagina davvero nell'approccio passando dall'emergenza alla prevenzione. agricola comune (PAC) fino al 2020 ci dà l'occasione di modulare dal punto di vista nazionale le nuove politiche specifiche; questo è uno dei grandi temi che l'Italia dovrà mettere al primo posto proprio nei piani nazionali delle politiche agricole. Per l'agricoltore questo approccio di emersione dei servizi può rappresentare un importante fattore di valorizzazione, un nuovo corso nel mestiere dell'imprenditore agricolo. se nell'economia tradizionale altro non era che un'attività sottintesa e invisibile della produzione di alimenti, ora può emergere come servizio specifico di conservazione ambientale, di consolidamento dei versanti; così l'azienda agricola, singola o associata, può diventare uno degli interlocutori principe delle politiche di manutenzione dei versanti, della regimazione delle acque. A mio avviso, se davvero vogliamo parlare di una strategia della manutenzione diffusa e imponente che voglia essere efficace, bisogna saper ricercare nuovi soggetti della manutenzione. Si tratta di una strategia che potrebbe innescare una modernizzazione importante del settore agricolo, nuove conoscenze e nuove capacità dell'imprenditore agricolo, niente che assomigli all'assistenzialismo e al sostegno al reddito a prescindere, ma misurazione delle azioni, competenze, nuova occupazione di qualità, criteri e parametri definiti. Occorre una nuova concezione del governo del territorio, in cui erosione del suolo, scarsità dell'acqua e devastazione da troppa acqua siano temi non marginali, ma centrali, una sorta di autogoverno consapevole del territorio in una responsabilità condivisa tra sistema pubblico e impresa agricola, una nuova concezione della ruralità come rivitalizzazione dei valori territoriali ed etici, perché parliamo di responsabilità verso le generazioni future. se è vero che le crisi più profonde sono determinanti per cambiamenti coraggiosi, anche se questo è un momento veramente difficile, è possibile indicare nuove scelte, evidenziare una nuova centralità dell'agricoltura e questa ne è la premessa. Non è più una questione settoriale, ma qualcosa che appartiene a tutta la società civile. Oggi emerge la richiesta di una classe dirigente politica che abbia occhi per vedere tutto questo.*(Applausi

Io però vorrei porre l'attenzione su qualcosa di diverso. C'è un professore, un geologo napoletano, che dice che il dissesto idrogeologico è indubbiamente figlio del dissesto ideologico: siamo stati cicale quando avremmo dovuto essere formiche; abbiamo dissipato un capitale enorme. E ora, se chiedessimo alla formica di Esopo cosa fare, ci risponderebbe. «Hai cantato? E allora adesso balla!».

amministratori spendendo solo 2 miliardi in 20 anni per la manutenzione del suolo, per spendere poi in realtà ben oltre 200 miliardi per arginare le emergenze. Siamo stati furbi, no? Siamo stati bravi amministratori o piuttosto bravi finanziatori di qualcuno? Perché questi ingenti stanziamenti sono serviti soprattutto per il funzionamento dell'ingombrante macchina emergenziale.

non più di 40 miliardi di euro. Quindi ne avremmo risparmiati ben 160: ripeto, avremmo risparmiato 160 miliardi di euro. Allora sì che avremmo potuto dirci dei buoni amministratori del bene comune, non del bene particolare di alcuni. Naturalmente non abbiamo sbagliato solo a non investire, abbiamo sbagliato a pianificare. Lo abbiamo detto tutti, lo ha ricordato soprattutto il mio collega. Abbiamo lasciato che i vincoli idrogeologici e i piani per l'assetto idrogeologico (PAI) non venissero rispettati; abbiamo permesso che la cementificazione selvaggia arrivasse - con opere abusive o parabusive - a mettere a rischio la vita della gente, chiudendo gli occhi e prendendo mazzette, come se fosse un danno da poco. Facciamo sempre questo errore: non guardiamo la cosa nel dato complessivo. Abbiamo la vista corta, noi italiani, e non vediamo oltre il nostro naso. La nostra penisola è caratterizzata dall'avere un territorio particolarmente fragile, per la sua relativa giovinezza, con uno sviluppo costiero estesissimo, che in buona parte già è interessato da un crescente grado di erosione. Ed è anche un territorio generalmente sismico, perché soggetto alla tettonica delle placche. Negli ultimi anni - ho sentito dire - i fenomeni naturali che hanno generato morte sono stati 237, con quasi 2.000 vittime. Ricordiamo il Vajont, la Valtellina, il Piemonte, il Sarno (nel 1998). Quindi il nostro è un territorio particolare e prezioso, che avremmo dovuto preservare; non l'abbiamo fatto e non lo stiamo facendo ancora. Non lo sta facendo questa maggioranza con i progetti che ha in atto. Cosa stiamo facendo invece? Pensiamo di risanare l'Italia trivellando il Paese in lungo e in largo per i folli deliri di un'Italia petrolizzata, alla ricerca spasmodica del petrolio cattivo, del petrolio del fondo del barile? Non si può certo pensare di risanare l'Italia come se qui non ci vivesse nessuno, realizzando metanodotti dall'Algeria, corridoi sud dell'Adriatico, rigassificatori, raddoppiando l'estrazione di idrocarburi; come se in questo Paese non ci vivesse nessuno, ed è invece un Paese troppo antropizzato e malamente urbanizzato, disboscando, cementificando gli alberi, artificializzando i corsi d'acqua e gettandovici finanche i rifiuti. Tutto questo ha generato un cambio di rotta, ha aperto gli occhi sulla necessità di cambiare strategia? No. La misura è colma. Mentre noi siamo qui tutti a parlare e a chiedere al Governo di impegnarsi per uno sforzo straordinario (tranne qualcuno che parla di assicurazioni private, questo mi ha un po' sconcertata), per la preservazione del territorio, al fine di mantenerlo in un equilibrio idrogeologico, questo stesso Governo è impegnato direttamente indirettamente in un'impressionante ed inarrestabile opera di devastazione del territorio, realizzando e progettando grandi opere inutili. Ma lo vogliamo capire una buona volta che l'unica vera grande opera strategica del nostro Paese deve essere la messa in sicurezza del territorio e la sua bonifica? salvaguardare le acque dall'inquinamento e proteggere le popolazioni dalle acque, per citare il mio collega Cioffi, recuperare strutturalmente i nostri beni primari, le nostre vere ricchezze, ricchezze, i nostri patrimoni, che al contrario continuiamo a saccheggiare come se non se ne dovesse vedere mai la fine. Ma la fine è vicina. Abbiamo saccheggiato, dilapidato, svenduto e ci accingiamo ancora a farlo. Proteste inascoltate contro le grandi opere inutili si moltiplicano in tutto il Paese. La storica e stoica resistenza delle comunità in Val Susa è nota a tutti e ne parlano anche gli intellettuali come De Luca, che la assimila ad un paese occupato da un esercito straniero. Ed è vero, visto che bisogna consegnare i

ve ne vorrei riportare uno segnalatomi dal mio collega Enrico Cappelletti, oggetto di una recente interrogazione del Movimento 5 Stelle al Ministero dell'ambiente. La città di Vicenza va sott'acqua più o meno ogni anno. Ogni volta ci stupiamo di fronte alle vittime e ai danni, ma non ne traiamo alcuna lezione perché dimentichiamo che all'origine dei guai sono sempre l'opera dell'uomo, la cementificazione dei territori, il disboscamento lungo i fiumi e la mancanza di una manutenzione geologico-idraulica del territorio. All'origine degli allagamenti di Vicenza vi è la recentissima realizzazione in città di una imponente speculazione edilizia di oltre 100.000 metri quadri (il nuovo tribunale di Vicenza sorto a Borgo Berga, ribattezzato 1'ecomostro di Vicenza) e del complesso edilizio adiacente in costruzione, tutto a ridosso degli argini dei fiumi Retrone e Bacchiglione, in totale violazione del rispetto del vincolo dei 10 metri di distanza dalle sponde dei fiumi medesimi. Cappelletti dice: «Qui ci sono responsabilità politiche superiori rispetto a quelle civili e penali, responsabilità delle due giunte di colore diverso che hanno governato nell'ultimo decennio e che hanno portato in una delle zone più pregiate della città, una zona dove è difficile costruire una veranda in terrazza per un comune cittadino, questa schifezza sorta sopra un terreno contaminato da fanghi e petrolio, una discarica di prodotti industriali non bonificata». «il peccato originale di questo ecomostro sono i 25 milioni di euro stanziati dal Governo Berlusconi per costruirlo, su un terreno che era di proprietà dell'impero economico e finanziario proprio della famiglia del pregiudicato più famoso d'Italia, Silvio Berlusconi. Insomma, un enorme conflitto di interessi». rivolge un augurio alla città: «La città tedesca di Dresda è stata estromessa dalle città patrimonio dell'UNESCO perché ha costruito un ponte; il mio auspicio è che non passi un funzionario dell'UNESCO anche a Vicenza». Fermare questa imponente operazione di cementificazione in corso si può ancora fare. Colleghi, occorrono scelte coraggiose - e non solo parole rivolte a rivedere e limitare fortemente il consumo del suolo, ma scelte necessarie per prevenire un ulteriore, drammatico ed inevitabile dissesto. Fermiamo il cemento prima che il cemento fermi tutti noi.

come è noto i rischi idrogeologici nel nostro Paese sono alquanto diffusi e in continuo divenire: rischi che, in un contesto così antropizzato qual è il territorio italiano, hanno prodotto nel tempo più di 150.000 vittime ed uno spreco di risorse economiche paragonabile a diverse manovre finanziarie. Diventa perciò doveroso affrontare una severa e rigorosa politica di previsione e di prevenzione, che deve necessariamente rendere partecipi tutte le strutture scientifiche, tecniche ed istituzionali del Paese: dall'università, alla ricerca, dal mondo professionale a quello amministrativo, con le Regioni, le Province autonome e gli enti locali Occorre, quindi, attivare una corretta gestione del territorio verso lo sviluppo ecocompatibile e la sicurezza ambientale, riducendo drasticamente o, comunque, riportando entro limiti accettabili gli effetti deleteri derivanti dalle pericolosità naturali, quale è appunto il dissesto idrogeologico. Il dissesto idrogeologico è purtroppo diffuso quasi in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, producendo in termini di vite umane e di danneggiamenti prezzi ancora più elevati di quelli causati dagli eventi tellurici e dalle eruzioni vulcaniche. Secondo l'Istituto di ricerca e protezione idrogeologica del CNR, nel Paese dal 1960 ad oggi ci sono stati 1.443 avvenimenti inclementi tra frane, crolli e inondazioni, con 4.122 morti e 2.850 feriti. Di fatto, in Italia, quasi l'82 per cento ha problemi di rischi idrogeologici: infatti, 1.700 di essi sono a rischi frana, 1.285 a rischio alluvione e addirittura 2.596 corrono entrambi i pericoli, con la conseguenza - ad essere precisi - che in cinquant'anni nel Paese si sono censite qualcosa come 500.000 frane.

Negli ultimi quattro anni, gli investimenti del Ministero dell'ambiente destinati a tenere sotto controllo il rischio idrogeologico sono stati quasi azzerati. un taglio ingiusto e non ne capiamo il motivo. Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, crediamo davvero di risparmiare tagliando i fondi per la prevenzione dei rischi idrogeologici? Questa è la domanda che ci dobbiamo porre. Io penso proprio di no, perché è certificato che lo Stato, in caso di eventi disastrosi, rischia di spendere almeno dieci volte di più, perché, in mancanza di interventi mirati, i costi per la riparazione dei danni e per la rimozione dei flussi fangosi sono enormi. resto già successa per le alluvioni del Veneto, della Toscana, delle Marche e della Campania, per le frane in Sicilia o, ancora, per gli eventi alluvionali dei mesi scorsi nei territori dell'Emilia-Romagna e della Liguria.

Ciò nondimeno, c'è da denunciare che nel Paese, con un territorio allo sfascio dalle Alpi a Pantelleria, questi rischi vengono spesso ancora ignorati e trascurati dai responsabili della pianificazione territoriale, adducendo come giustificazione la loro fatalità, quando nei fatti gli eventi calamitosi si presentano sistematicamente ora in una Regione, ora nell'altra. Parlare, quindi, di imprevedibilità o di sorpresa geologica è da irresponsabili, proprio perché la difesa dai rischi e dai dissesti idrogeologici si impone in termini di previsione e di prevenzione. In Italia purtroppo manca ancora la cultura del recupero ambientale, che di fatto si traduce nella previsione e nella prevenzione. Non ci si rende conto che il Paese è ad altissimo rischio e necessita di essere curato ed attenzionato perché è oltremodo soggetto a fragilità strutturali. Da noi si dovrebbero imporre prudenza ed intelligenza urbanistica, bloccando le continue deroghe alla normativa urbanistica, le costruzioni abusive ed invasive, la cementificazione selvaggia e la predazione inconsulta del territorio. Si dovrebbe invece investire, con adeguate forme di pianificazione territoriale, sulle opere di prevenzione e soprattutto sull'agricoltura, la quale non può essere abbandonata, perché, unitamente ai boschi ed alle pinete, presidia e cura il territorio ed il suo assetto vegetazionale e, come tale, costituisce la vera paladina per la lotta al dissesto ed al rischio idrogeologico, al degrado ed ai cambiamenti climatici. Vi è perciò l'obbligo per il Governo ed il Parlamento di adottare politiche di riqualificazione in favore dell'agricoltura e del suo valore strategico come presidio fondamentale ed unico per il consolidamento e la manutenzione straordinaria del territorio e dell'ambiente, così da contrastare la desertificazione delle colline e delle montagne per il ripetersi di episodi calamitosi ed emergenziali sempre più gravi e difficilmente risolvibili con l'abbandono della campagna e degli spazi rurali, soprattutto da parte delle giovani generazioni. Risulta, dunque, evidente che gli interventi integrati e di prevenzione ambientale, unitamente ai piani di messa in sicurezza del territorio, sono i soli che possano interrompere nel futuro le criticità idrogeologiche. Per non parlare, poi, dei terremoti o delle eruzioni vulcaniche, fenomenologie del resto alquanto presenti nella nostra penisola. Nel nostro Paese siamo sempre in ritardo sui temi di politica ambientale. Nel settembre 2012, dopo il rovinoso crollo di una delle passeggiate più belle del mondo, la via dell'amore, alle Cinque Terre, il Ministro dell'ambiente di allora, Clini, dichiarò che si sarebbe fatto immediatamente un piano nazionale di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio. Purtroppo, dopo un anno, siamo ancora in attesa. del problema sarebbe opportuno rilanciare, con forme di partecipazione attiva soprattutto nelle scuole e tra i giovani, Bisogna rendersi conto che un piano di riduzione e gestione dei rischi idrogeologici costituisce uno straordinario strumento di rilancio economico ed occupazionale e come tale deve essere affrontato, superando l'approccio agli interventi *una tantum* o di somma urgenza che - progettati sulla base dell'emotività del momento e, aggiungerei, di interessi particolari - non sempre riescono a risolvere i gravi problemi connessi ai dissesti idrogeologici dei suoli; problemi così critici che, talune volte, costituiscono una seria minaccia per la perdita delle naturalità e delle biodiversità. Purtroppo, signora Presidente, ci si ricorda di intervenire con programmi integrati di difesa e manutenzione idrogeologica del territorio unitamente alla riqualificazione ambientale soltanto al prodursi delle emergenze

perché ha voluto tratteggiare, esattamente come hanno fatto la collega Nugnes, i colleghi del Gruppo del Partito Democratico ed altri che li hanno preceduti, la necessità e l'urgenza di lavorare sul tema

il collega Vaccari, di portare avanti con determinazione progetti di legge che possano effettivamente riportare l'Italia nell'alveo

e quindi mi rivolgo, anche a lui quando dico che abbiamo opportunità straordinarie, di cui sarebbe opportuno che prendessimo atto quando parliamo del grave *deficit* e del grave ritardo che vive il nostro Paese su queste tematiche.

all'analisi dell'esistente riusciremo a produrre (lo spero e me lo auguro), con un intendimento che mi pare comune e collettivo, un'inversione di tendenza rispetto al tema dei corpi idrici.

fin da subito, a fare ragionamenti molto concreti, come si conviene a chi deve trovare risorse per risolvere i problemi.

nelle disponibilità del patrimonio europeo, restituendole di fatto ad una casa comune che ce le offriva per migliorare la nostra qualità ambientale.

locali possano effettivamente avere le risorse necessarie per mettere in ordine un territorio che è stato disordinatamente organizzato e che paga lo scotto di questa cattiva organizzazione. Quando parliamo di grandi opere, non diciamo mai che cosa esse producono in termini di occupazione: produce da 10.000 a 20.000 posti di lavoro per ogni miliardo investito. Si tratta di una quantità enorme perché si moltiplicano i posti di lavoro

cosa fondamentale per riuscire a gestire in maniera oculata e produttiva il territorio. Utilizziamo, dunque, i fondi comunitari che ci vengono messi a disposizione dalla PAC per

è in corso un lavoro tra i Gruppi, che spero possa avere buon esito, per la formulazione di un ordine del giorno unitario, di convergenza, in sostituzione delle singole mozioni presentate dai Gruppi.